Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, il contenuto dell'interrogazione, cui spero abbia già ricevuto il testo, è inerente agli investimenti per la riqualificazione del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Come lei sa, signor Ministro, questo è un argomento particolarmente sensibile nella nostra Regione, rispetto

mitigare gli effetti del sisma sulle strutture sanitarie e di ridurre il rischio sismico per tutte le strutture sanitarie abruzzesi, emerso inequivocabilmente in occasione del terremoto del 6 aprile

nell'ottica di ridurre i costi a regime della gestione delle strutture sanitarie, è logico che la scelta di costruire alcuni

ci dicono che le cose non vanno esattamente come da programma del Governo e del legislatore. Per quel che riguarda l'Abruzzo, dopo un lungo periodo di commissariamento, per così dire tecnico,

l'atto più significativo approvato dal commissario Chiodi è stato quello del cosiddetto programma operativo, così come previsto dall'articolo 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009,

a modo di vedere di chi ha voluto e impostato quel lavoro, ad ottenere risparmi e, in via teorica, più efficienza.

il Servizio sanitario regionale è tuttora caratterizzato, oltre che da incompetenza, da situazioni di diffusa illegalità, con fenomeni di corruzione (senza precisare quali). I dati finanziari sono tuttora

Cosa sta facendo il Governo per monitorare la situazione della sanità abruzzese? Cosa sta facendo per rimuovere

viene testimoniato dall'aumento della mobilità all'interno della Regione Abruzzo e dalle evidenti difficoltà riscontrate nei presidi ospedalieri.

Lei sa che è iniziata nel settembre 2008 con un commissario inviato dal Governo Berlusconi e continua con il commissariamento del presidente della giunta regionale, iniziato nel dicembre 2009. Entrambi i commissari avevano avuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri la delibera di nomina per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.

2007-2009, che è l'unico approvato dalla Regione Abruzzo e sottoscritto insieme al Governo, oppure sta

Se sta applicando il piano di rientro precedente, lo sta facendo con una discrezionalità che esula dalle competenze e dalle prerogative di un commissario *ad acta*. Cito alcuni esempi: nella ricontrattazione dei tetti di spesa con gli erogatori della sanità privata ha ottenuto risparmi di gran lunga inferiori rispetto agli obiettivi di piano, a vantaggio quindi delle strutture sanitarie private;

il Consiglio di Stato dichiarando che la riconversione di uno di questi ospedali (quello di Guardiagrele) non poteva avvenire se non si prevedevano adeguate misure alternative.

Se viceversa si tratta di un nuovo piano di rientro, signor Ministro, in qualità di rappresentante del Governo abbia la bontà di dire al commissario *ad acta* che un piano di rientro nuovo viene approvato secondo le procedure dell'intesa Stato-Regioni del dicembre 2009, e quindi approvato dalla Regione approvato dal tavolo di monitoraggio e dalla Conferenza Stato-Regioni, e poi approvato dal Consiglio dei ministri. Di certo non può essere un piano di rientro personale, autoreferenziale, all'insaputa dell'Abruzzo.

le procedure e le modalità di utilizzo di tali somme nell'ambito di un affiancamento costante. La procedura prevede che venga definito uno specifico accordo di programma, programma, comprensivo di un protocollo d'intesa e di un documento programmatico, nel quale sono definiti gli interventi da porre in essere in coerenza e in attuazione del piano di razionalizzazione e riqualificazione della rete territoriale e ospedaliera. I relativi documenti sono in fase avanzata di stesura. Pertanto, si conferma che, in presenza di un documento programmatico definito

Dalla data di insediamento del presidente Chiodi a commissario, la Regione ha fatto notevoli passi avanti sia in termini di programmazione che di contenimento dei costi. Per quanto riguarda questi ultimi, per l'anno 2010 si profila un disavanzo non coperto al netto degli ammortamenti non sterilizzati di soli 5 milioni milioni di euro, con un miglioramento deciso rispetto al 2007, in cui si era registrato un disavanzo non coperto di 76 milioni di euro. operativo elaborato dalla gestione commissariale, con il supporto e l'affiancamento del Ministero della salute e dell'AGENAS, interviene sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, sulla razionalizzazione dell'assistenza territoriale, sulla revisione della rete di emergenza‑urgenza, sulla razionalizzazione della rete dei laboratori pubblici e sul contenimento della spesa farmaceutica. Attualmente, i tavoli di monitoraggio certificano che si stanno attuando le azioni previste. Nei tavoli di monitoraggio è stata infatti valutata positivamente la manovra di riassetto strutturale ospedaliero, soprattutto per quanto attiene al contenimento del numero delle unità operative complesse e al piano di riorganizzazione della rete laboratoristica. la Regione ha provveduto all'approvazione di tre importanti documenti di programmazione ospedaliera. Il primo concerne la metodologia di definizione del fabbisogno di prestazioni ospedaliere e dei posti letto correlati. Vorrei che si noti la *consecutio* anche logica dei vari documenti approvati

In tema di riduzione delle prestazioni inappropriate, la Regione ha predisposto uno schema di delibera commissariale, cioè il piano regionale per la riduzione riduzione delle prestazioni inappropriate, che prevede il trasferimento dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza, per una quota, in regime di *day hospital* e, per una quota, direttamente in regime ambulatoriale.

come si vede, i dati dimostrano che effettivamente c'è un'attività concreta per realizzare il piano di rientro. la gestione commissariale ha svolto il procedimento previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1993 in materia di programmazione assistenziale. Infatti sono state definite le linee negoziali per regolamentare i rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate e dalle case di cura private, nonché le prestazioni rese da studi medici, nel rispetto dei tetti di spesa 2010. L'insieme di questi elementi evidenzia che la gestione commissariale, pur in presenza di straordinarie difficoltà di contesto legate alla gestione emergenziale del *post*-terremoto (che vanno tenute in considerazione), sta adempiendo, per quanto attiene alla certificazione dei tavoli tecnici di monitoraggio, al mandato conferito dal Consiglio dei ministri per l'attuazione del piano di rientro e sta anche adottando delle procedure di programmazione e di gestione regionale basate su metodologie e criteri trasparenti che siano in grado, da un lato, di qualificare l'assistenza sanitaria e, dall'altro, di «blindare»

la salute (NAS) per il potenziamento dell'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio delle strutture sanitarie regionali. Questo processo di sostanziale recupero dell'equilibrio di bilancio e di avvio del percorso di razionalizzazione e qualificazione della rete sanitaria e sociosanitaria è stato gravato da un pesante elemento di difficoltà ascrivibile a responsabilità dei governi regionali che hanno preceduto la presidenza Chiodi. Infatti, nel corso delle verifiche effettuate nell'anno 2010, è emerso che la Regione Abruzzo, a suo tempo, con le precedenti gestioni ha dirottato verso altri settori della spesa regionale cospicue risorse del servizio sanitario regionale, per il finanziamento della spesa corrente con riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006, per complessivi 331 milioni di euro, con la conseguenza che, riportando a nuovo la corrispondente passività e sommando ad essa i disavanzi non coperti negli anni 2007 e 2008 per un importo di 81 milioni di euro, l'attuale gestione sanitaria della Regione Abruzzo si trova ad essere ancora gravata da un disavanzo di ben 412 milioni A fronte di tale situazione provocata dalle precedenti gestioni, l'attuale gestione commissariale ha adottato i decreti n. 3 del 2008, n. 25 del 2009, n. 26 del 2009 e n. 27 del 2009, con cui ha reintegrato le risorse del servizio sanitario regionale per circa 115 115 milioni di euro. Per la rimanente parte da coprire dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti che saranno concertati con i Ministeri affiancanti. PRESIDENTE. Hanno

quanto siano importanti le risorse per la ristrutturazione delle strutture ospedaliere, sia per il servizio sia per l'efficienza della macchina sanitaria abruzzese. Ringrazio inoltre il Ministro per aver fatto, anche se sinteticamente, chiarezza sul percorso che in questi anni sta affrontando la Regione Abruzzo e in particolare il commissario alla sanità Gianni Chiodi. Signora Presidente, a differenza del senatore Tancredi, mi ritengo totalmente insoddisfatto, perché a tutti i quesiti che abbiamo posto non è stata data risposta. risposta. Il programma operativo approvato è stato sanzionato dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale come atto illegittimo. Il Governo non può ignorare questo dato sulla base del quale si sarebbero verificati i fatti esposti dal Ministro. Abbiamo chiesto al Ministro e continueremo a chiedere perché

con atti palesemente illegittimi e che stanno sfasciando la sanità Presidente, mi ritengo parzialmente soddisfatta, nel senso che sicuramente il Ministro non è riuscito a darci un censimento definitivo dello

prendo atto che in Abruzzo esiste un solo piano di rientro, che era quello vigente al momento della nomina del commissario *ad acta.* Tutto il resto sono variazioni che godono di una discrezionalità e che esulano dai compiti di un commissario. I suoi dati, signor

è priva della contestuale costruzione di una rete di emergenza territoriale di medicina dei servizi e di medicina del territorio. E per quanto riguarda

sanitario nazionale, il commissario dichiara di aver bisogno di un anno di tempo, lo chiede alle procure e ai TAR (mi è nuovo che le procure partecipino alla politica sanitaria), e lo chiede perché ha bisogno di una tolleranza in una situazione di non perfetta legalità.

signor Ministro, lei sa perfettamente, come ha detto oggi in Commissione sanità, che non ci possiamo più permettere una «sanità del campanile». Bisogna avere il coraggio e la volontà politica e amministrativa di ristrutturare il sistema sanitario, specialmente in quelle Regioni che sono poste sotto attenzione per il rientro della spesa sanitaria. sanitaria. Vivo nel Lazio, che è una di quelle Regioni, e quindi so perfettamente cosa vuol dire accorpare reparti, riorganizzare il servizio, dare risposte adeguate sapendo di dover tagliare tutti quei rami secchi che non producono nel sistema sanitario né capacità professionale né tanto meno attenzione nei riguardi degli assistiti. Per questo le pongo la seguente domanda: non ritiene che la chiusura del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Crotone rientri nel contesto generale della riorganizzazione e della risposta organizzativa che anche nel territorio calabrese va data

merita da un lato sicuramente l'abbattimento del tono polemico del dibattito, ma dall'altro anche una riflessione particolare ed approfondita in concomitanza con il piano di rientro dal *deficit*, di cui è titolare, su delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio scorso, il presidente della Regione. Indubbiamente è essenziale anche una rivisitazione del sistema ed una coerente razionalizzazione dei presidi ospedalieri, ma ciò sicuramente non può incidere in maniera drammatica su alcuni contesti. Mi riferisco specificamente all'abbattimento del reparto di infettivologia dell'ospedale di Crotone che, per altro, ha operato sicuramente in maniera esemplare, dando una grossa tranquillità ai pazienti calabresi di quell'area. Vorrei sottoporre alla sua attenzione, signor Ministro, due contesti: due contesti: da un lato, abbiamo una struttura che ha operato molto bene a beneficio dei cittadini calabresi; dall'altro, abbiamo una grossa preoccupazione sull'abbattimento di questo reparto, in riferimento anche ad una presenza

coscienti della necessità di un piano di rientro che rimetta in sesto la sanità calabrese. Qualche giorno fa, però, anche il Comitato parlamentare Schengen si è recato presso il centro di accoglienza Sant'Anna di Crotone,

in una realtà così importante - dobbiamo ricordare che in questi giorni sono presenti più di 1.200 immigrati stranieri con grosse problematiche di salute

quanto sono in aumento tutte quelle patologie infettive tipo la tubercolosi e l'HIV che in tali realtà

chiediamo che esso non venga fatto soltanto sulla carta, ma tenendo presenti le necessità oggettive di efficienza e di servizio per i cittadini sia stranieri che calabresi.

I parametri previsti dall'AGENAS, che sono stati di supporto alla predisposizione del Piano di rientro della Regione Calabria, determinano una struttura complessa di malattie infettive per ogni DEA di secondo livello (*Hub*); i

Quindi, in Calabria sono previste tre strutture complesse di tale disciplina (primariati): una a Catanzaro, una a Cosenza e una a Reggio Calabria, tutte sedi di DEA di secondo livello. La Regione può, laddove vi siano esigenze specifiche nel settore della patologia infettiva, prevedere strutture semplici di malattie infettive in qualche DEA di primo livello (*Spoke*) all'interno dei dipartimenti di area medica. Comunque, il piano di riordino deliberato dalla Regione Calabria non è stato ancora approvato dai tavoli di monitoraggio e quando nel tavolo di affiancamento del Ministero della salute ed AGENAS alla Regione sarà concordata la proposta definitiva della rete ospedaliera, potrà anche essere presa in considerazione una diversa articolazione della rete di malattie infettive, tenendo sempre conto delle compatibilità economiche sottese al piano di rientro. effetti, onorevoli senatori, i recenti sbarchi di immigrati stranieri cambiano il quadro e credo che la questione potrà, anzi ritengo dovrà, essere riesaminata proprio alla luce della massiva presenza di immigrati

delle risposte date poc'anzi dal Ministro, in quanto le tre DEA di secondo livello da lui citate sono sufficienti, a mio avviso, per la Regione Calabria.

portare dei pazienti da un territorio all'altro sicuramente costa di più. Si tenga presente, e con ciò voglio rispondere al senatore Gramazio, che questa non è un'emergenza:

stabile, che ci costringe a chiedere la presenza di un reparto di malattie infettive e di dermatologia, perché altrimenti questi pazienti dovrebbero essere ricoverati in un reparto di medicina interna,

finestra"). Ringrazio il ministro della salute, professor Fazio, per la disponibilità e dichiaro concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.